La Commissioni e i due relatori hanno esaminato il testo articolo per articolo, emendamento per emendamento, proprio per cercare di portare alla discussione dell'Assemblea un testo rafforzato rispetto agli obiettivi iniziali del decreto-legge. Questo è un provvedimento che ha l'ambizione di rilanciare l'economia del Mezzogiorno e di ridurre significativamente il profondo e sedimentato *gap* tra Nord e Sud del nostro Paese, il tutto con misure tese a rafforzare e a consolidare la crescita e a scoraggiare il triste fenomeno dell'emigrazione verso Nord della forza lavoro, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei giovani. Non a caso già all'articolo 1 viene introdotta la misura, che tutti ormai conosciamo, denominata «Resto al Sud». Si tratta dell'opportunità per i giovani *under* 35 di avviare un'attività imprenditoriale nelle Regioni del Mezzogiorno a condizioni particolarmente vantaggiose, ossia con un finanziamento che è stato esteso, grazie al lavoro in Commissione, fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 35 per cento e il restante 65 per cento attraverso un prestito a tasso zero da restituire in otto anni. Un'altra modifica importante ha riguardato l'ampliamento dell'applicabilità della stessa misura ai servizi turistici, alla pesca e all'acquacoltura.

giusta e corretta per rilanciare il Sud, creare occupazione e nuove prospettive per i giovani e offrire un'opportunità a chi oggi rimane ai margini dell'occupazione, decidendo

ossia le zone in cui le imprese già insediate o che si insedieranno godranno di semplificazioni amministrativo-burocratiche e fiscali, tra cui certamente il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, nel limite massimo di 50 milioni di euro. Le imprese dovranno mantenere le attività nelle Zone economiche speciali per almeno sette anni previsto nel decreto-legge - successivi al completamento dell'investimento oggetto dell'agevolazione. Lo scopo delle ZES è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese e saranno concentrate nelle aree portuali collegate alla rete

Grazie al lavoro svolto in Commissione è stata data la possibilità alle Regioni interessate di presentare una o al massimo due proposte di istituzione di ZES, quando siano presenti più aree portuali collegate alla rete transeuropea dei trasporti. Per quanto riguarda invece le Regioni che non hanno tali aree portuali sarà possibile presentare istanza in forma associativa, se contigue, o in associazione con un'area portuale che abbia le caratteristiche previste. Le ZES saranno attivate su richiesta delle Regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro *governance*. Le diverse esperienze di ZES saranno messe a sistema, in un'ottica di sviluppo strategico, attraverso il coordinamento generale garantito a livello centrale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 12 sono stati approvati dalla Commissione degli emendamenti volti a trovare i giusti equilibri nei criteri di riparto del fondo università statali:

le esigenze di tutela degli atenei del Sud che operano in contesti economici e sociali svantaggiati. All'articolo 14 è stata inserita un'ulteriore proroga di due mesi dei termini per la consegna di beni strumentali funzionali ai processi di digitalizzazione

Con un emendamento del Governo, infatti, è stato previsto all'articolo 423-*bis* del codice penale, ferme restando le pene vigenti in materia di incendio doloso, che, nel caso in cui il proprietario bruci per qualsiasi ragione il proprio terreno, quest'ultimo sarà oggetto di confisca a beneficio del Comune in cui il terreno è situato. Inoltre, la novella stabilisce che se il proprietario del terreno bruciato è stato vittima di estorsione compiuta attraverso la violenza o la minaccia di commissione del reato di incendio doloso, il terreno incendiato potrà avere, sempre nel rispetto degli strumenti e disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, anche una diversa destinazione d'uso. Si tratta di misure efficaci per contrastare in maniera concreta un reato grave e dilagante.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

tale sistema sarebbe utile anche per decongestionare i centri storici delle nostre città dall'assedio di veicoli commerciali. nei centri storici delle città di Palermo e Matera solo se questi mezzi saranno costantemente e tempestivamente monitorati e controllati dalla nostra piattaforma digitale. Il rilancio degli investimenti ha puntato in particolare sui *driver* dello sviluppo, che sono direttrici d'intervento prioritarie, motori che possono far diventare il Sud un'opportunità di sviluppo per l'Italia in esame reca un insieme di interventi utili, importanti, a mio e a nostro avviso anche improcrastinabili,

a destinare 90 milioni alla ristrutturazione e messa in sicurezza dei tribunali del che qualcuno possa sostenere che si tratta di un provvedimento destinato a una parte del nostro Paese piuttosto che a un'altra,

il completamento delle altre parti che devono essere portate a conoscenza dell'Assemblea, ringraziando ancora tutti i componenti della Commissione, il presidente Tonini, ma soprattutto il Governo nella persona del ministro De Vincenti, che con pazienza

Mi chiedo cosa siano una politica e un'azione di Governo, se non un insieme di misure e di interventi all'interno di una visione. visione. La concretezza del provvedimento che ci accingiamo ad esaminare corrisponde a un altro significativo pezzo di una rinnovata politica per il Mezzogiorno che questo Governo, il Governo Gentiloni ha inteso consolidare, in continuità con le misure avviate negli anni passati dal Governo Renzi. Una politica per il Mezzogiorno che in questi ultimi due anni ha preso forma, provando finalmente a mettere a sistema la finalizzazione delle risorse pubbliche comunitarie e nazionali, risorse che in realtà - diciamoci la verità - non sono mai mancate, ma che hanno vissuto spesso, negli anni e nei decenti passati, gestioni dispersive e poco incisive. ancora, accanto a una finalizzazione organica di queste risorse, in questi anni finalmente è stata messa in campo una *governance* unitaria e al tempo stesso integrata tra Governo nazionale, Regioni e comunità locali.

con il contratto istituzionale di sviluppo. Si è trattato di un lavoro per nulla semplice, che ha coinvolto Regioni e comunità locali nell'individuazione delle priorità nel campo degli interventi infrastrutturali, nonché di carattere industriale e sociale, che attiverà a regime circa 90 miliardi di risorse nei prossimi sei anni e che già ad oggi ha attivato - sicuramente il ministro De Vincenti potrà essere più preciso - circa 700 cantieri, per circa 7 miliardi di euro di investimenti. Si tratta di un lavoro impegnativo, che proprio il ministro Claudio De Vincenti ha coordinato con straordinaria generosità e con grande impegno. Lo voglio quindi ringraziare

trovando anche una sintesi più avanzata rispetto al testo con cui il decreto-legge è giunto alle Camere. Una disponibilità grazie alla quale abbiamo potuto lavorare, collaborare, condividere; uno sforzo verso l'ulteriore rafforzamento delle misure che qualificano il provvedimento al nostro esame. Un altro pezzo di questa rinnovata politica che fa dell'attenzione verso quella parte del Paese una questione prioritaria per l'intero Governo e per l'intero Paese.

ci ha portato ad esaminare oltre 800 emendamenti e ad approvarne oltre 100 provenienti da tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Vi è in questo numero

va collocato un provvedimento come quello che stiamo esaminando, che ha affrontato alcune mirate emergenze e priorità, ma soprattutto ha previsto una serie di misure finalizzate a favorire la crescita economica ed occupazionale del Mezzogiorno, a cominciare dalla misura «Resto al Sud» - ne ha parlato la senatrice Vicari - di cui ricorderò solo un aspetto. C'è tanta voglia da parte dei giovani del Mezzogiorno di mettersi in gioco, non solo per rimanere in quella parte del Paese,

la possibilità per le Regioni di cofinanziare queste misure e questi interventi ove le risorse nazionali non dovessero bastare. Ci abbiamo creduto talmente tanto che impegniamo anche le Regioni a dare il loro contributo. È una misura che poi si allarga al mondo dell'agricoltura e delle pesca, come abbiamo richiamato, in un *mix* di sperimentazioni di forme nuove di utilizzo delle opportunità che vengono

dei terreni incolti e degli immobili in disuso e abbandonati che, con una regia in capo agli enti locali, potranno costituire una sorta di banca cui attingere per sperimentare nuove modalità di fare impresa. La seconda misura che voglio richiamare - ne ha già parlato la collega Vicari - che a me sembra la seconda scommessa tra le più significative di questo provvedimento, è l'istituzione delle cosiddette Zone economiche speciali: una delle misure più importanti di questo provvedimento. Si tratta dell'istituzione di aree geograficamente delimitate, all'interno delle quali sono riconosciute alle imprese che vi si insediano condizioni favorevoli in termini economici, economici, di fiscalità, di snellimento di procedure e di facilitazioni amministrative. Secondo quanto abbiamo previsto nell'articolato, le ZES si concentreranno nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, alle quali verranno riservate agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta per il Mezzogiorno, oltre alla semplificazione di adempimenti e all'accelerazione dei termini procedimentali e per l'accesso alle infrastrutture esistenti. Delle Zone economiche speciali noi, in questo provvedimento, Delle Zone economiche speciali noi, in questo provvedimento, diamo finalmente una definizione giuridica, un contorno di regole che probabilmente potranno anche evolversi negli anni a venire; un quadro normativo cui attingere insieme alle Regioni, quindi di concerto con i territori, per delimitarne l'entità. Lo scopo è quello di sperimentare nel nostro Paese modalità di attrattività di alcune aree collegate alla portualità che ben hanno funzionato in altri Paesi in Europa e nel mondo, con un *mix* di crediti fiscali, di agevolazioni fiscali e di snellimenti procedurali. Abbiamo fatto anche un'altra scelta nel

e anche l'accademia, i centri studi, a cominciare dallo Svimez, che si sono molto cimentati sulla utilità di questa strumentazione per consolidare le potenzialità e metterle a regime nel Mezzogiorno d'Italia. d'Italia. In quegli studi, in quelle ricerche e anche in alcune posizioni politiche c'era l'idea che potessero bastare due, tre aree disseminate nel Mezzogiorno, ben concentrate. Si sono fatti anche nomi: Napoli, Gioia Tauro, Taranto. noi abbiamo fatto una riflessione diversa: forse è il caso di scommettere su una rete di Zone economiche speciali che accanto a questi tre grandi poli - le modifiche

per quanto riguarda sia nuovi investimenti sia la valorizzazione del patrimonio industriale, manifatturiero e della filiera logistica già esistente. Ciò consentirà ad alcune Regioni, quelle più grandi, di poter contare fino a due Zone economiche speciali - penso alla Puglia o alla Sicilia - e ad altre Regioni, dove non vi sono porti

Insomma, un'altra significativa scommessa che credo sia assolutamente da vincere e che sono certo il Mezzogiorno potrà cogliere al meglio. Altro tema è quello delle semplificazioni e ve ne sono diverse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

ad una misura che va nella direzione dello snellimento delle procedure per spendere le risorse dei cosiddetti patti per il Sud, di cui ho parlato all'inizio. Con questa norma di semplificazione, Regioni ed enti locali che adotteranno questi strumenti e che presenteranno progetti, con un semplice strumento di autocertificazione, potranno ottenere già prime anticipazioni. Altre semplificazioni intervengono nel settore dell'ambiente e dei rifiuti e degli *standard* degli *standard* finanziari tra Regioni ed enti locali. Sempre in tema di enti locali, voglio ricordare un intervento che guarda sì al Mezzogiorno,

destinati ad alleviare la sofferenza, la criticità finanziaria in cui vivono le Province e le Città metropolitane del nostro Paese, da assegnare alle funzioni fondamentali. Abbiamo ben chiaro come questi enti locali abbiano vissuto e stiano vivendo momenti di straordinaria difficoltà, che mettono in crisi la stessa capacità di erogare le funzioni fondamentali. In alcuni di questi enti si preannunciano addirittura rischi di dissesto finanziario e sono a rischio non solo le funzioni fondamentali, ma anche la stessa capacità di mantenere forza lavoro e funzioni.

La seconda misura è invece volta a consolidare il quadro normativo e giuridico che vincola le risorse rivenienti dalla confisca dei beni sequestrati ai Riva alla destinazione che era

al tema del risanamento ambientale, ma guardando a tutto il gruppo ILVA e, quindi, a tutti gli stabilimenti. Credo che l'idea della gestione commissariale e dello stesso Governo sia quella di destinare queste risorse agli altri stabilimenti del gruppo ILVA

il saldo sarà sicuramente positivo, in termini di ulteriori risorse e di attenzione a favore di questo nuovo meccanismo verso le università

Abbiamo raccolto le indicazioni venute da tutti i Gruppi,

per quanto riguarda gli interventi urgenti di smaltimento delle macerie che ancora insistono nell'area del cratere. Il provvedimento contiene inoltre norme di semplificazione e prevede il prolungamento dello stato di emergenza, l'allungamento dei tempi per la presentazione delle domande di indennizzo e l'eliminazione sembrerà un paradosso, ma c'è voluta una norma - della tassa di successione sulle case purtroppo distrutte dal sisma. Mi pare che anche in questo senso abbiamo fatto un buon lavoro, raccogliendo le indicazioni provenienti da tutti i Gruppi.

abbiamo ben chiaro come rimangano ancora debolezze e limiti irrisolti: pensiamo alle grandi infrastrutture, a cominciare dalle interconnessioni ferroviarie, alla necessità di consolidare al sistema produttivo, possiamo rivendicare con assoluta fermezza che in questi anni abbiamo invertito la tendenza, una tendenza che per troppo tempo ha visto un'attenzione verso il Mezzogiorno piena di parole e di impegni ma povera di atti e di politiche. Ora, lo possiamo ben dire, abbiamo una politica e finalmente atti e misure che vanno nella direzione di rilanciare e valorizzare per davvero le potenzialità del Mezzogiorno

Il decreto-legge in esame è il 71° provvedimento d'urgenza, se si sommano quelli del Governo Renzi e del Governo Gentiloni Continua, da parte dell'Esecutivo, un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, attraverso la quale si assiste al radicale e inaccettabile spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo. Il mio intervento non potrà quindi avere la caratteristica della novità rispetto agli interventi che in occasioni analoghe sono stati svolti da colleghi del mio Gruppo, ma questo non dipende da noi, bensì da un Governo che continua a replicare un *modus operandi* che umilia il Parlamento. Nello specifico, il decreto-legge reca misure a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, denominate «Resto al Sud»; interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere nel Mezzogiorno; istituzione di Zone economiche speciali; benefici fiscali e misure di semplificazione; disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo; valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo; disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria; misure in materia di costo *standard* per studente; disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA; misure in materia di assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali nel Mezzogiorno; misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale ed altre misure ancora. Tuttavia, a rendere immediatamente vana ogni velleità del provvedimento in esame viene la relazione tecnica, dalla quale si deduce che tutto il decreto-legge è fatto a saldo zero, nel senso che non stanzia neanche un centesimo aggiuntivo su quanto previsto per il 2017 e per il triennio 2018-2020. Dunque gli interventi previsti, che nelle intenzioni del Governo sono volti, da un lato, a superare il divario tra le Regioni del Sud d'Italia e il resto del Paese e, dall'altro, ad introdurre nuovi strumenti finalizzati alla crescita delle Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso misure per i giovani imprenditori, ci sembra non siano assolutamente sufficienti per raggiungere l'obiettivo economico che si propongono e, soprattutto, per determinare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Infatti, tali misure non solo potrebbero essere inserite in provvedimenti più razionali e coesi, ma addirittura, in alcuni casi, adottate con strumenti ordinari di razionalizzazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione, essendo l'unica fonte finanziaria da cui attingono. Invece, siamo, ancora una volta, in presenza di una stratificazione di disposizioni, di una modalità normativa scomposta e poco incisiva. Giova anche sottolineare che il carattere di omogeneità non può certo essere costituito dalla dalla destinazione degli interventi ad alcune aree del Mezzogiorno. Disomogeneità aggravata dagli emendamenti approvati in Commissione, tra i quali cito quello, secondo me veramente estraneo alla materia che deve essere oggetto di questo intervento, riguardante le norme di contrasto ai fenomeni degli incendi boschivi. Non è certamente in discussione la necessità di contrastare questo fenomeno,

nelcaso dei decreti-legge, che rappresentano una modalità straordinaria e non usuale con cui il Governo può legiferare, è necessaria l'ulteriore valutazione se in sede di conversione in legge le eventuali proposte di modificazione o di integrazione del testo contrastino con i principi di omogeneità delle disposizioni e di una loro necessità ed urgenza data da situazioni attuali e contingenti. Il provvedimento al nostro esame si somma ad un lungo elenco di analoghe iniziative legislative emanate dal Governo negli ultimi due anni, per i quali il possesso dei criteri di straordinaria necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, è residuale e l'omogeneità del testo risulta essere compromesso da disposizioni eterogenee che lo rendono disorganico. Inoltre, il provvedimento, proprio a causa del susseguirsi di disposizioni tra loro eterogenee, è oggettivamente carente di una sua linearità strutturale, nel senso che le materie trattate non risultano sequenziali e unite da un nesso. Giova ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale fonda da sempre i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo della omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge

costituisce «esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, Il provvedimento al nostro esame ancora una volta, evidenzia dunque storture che sono da considerarsi un palese abuso. in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per giustificare la necessità di emanare un decreto-legge. Oltretutto, si utilizza lo strumento del decreto-legge per riproporre una tipologia di misure vecchie, come quella dei finanziamenti a fondo perduto o a tasso zero, che hanno negli anni addietro ampiamente dimostrato di finire la propria portata nel momento in cui finiscono i finanziamenti a pioggia. Si tratta di misure già viste e sperimentate, che non riusciranno a far emergere iniziative imprenditoriali nuove, ma semplicemente a distribuire a pioggia somme a una platea di circa centomila giovani del Sud. Da ciò discende come vi sia un utilizzo politico improprio della decretazione d'urgenza, ravvisabile anche nel fatto che i provvedimenti emanati dall'Esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelli di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero che in termini di durata. Purtroppo dobbiamo constatare che qualsiasi iniziativa da parte del mio Gruppo volta a segnalare l'assenza dei principi di costituzionalità è risultata vana. Se, infatti, da una parte si registra la propensione del Governo ad un utilizzo della decretazione di urgenza per una celere realizzazione degli obiettivi della sua politica, cioè la decretazione di urgenza da intendersi come necessità e urgenza in relazione ai fini della realizzazione del programma di Governo, dall'altra parte si assiste ad una inopportuna condiscendenza da parte di questa Assemblea. Nel merito, va innanzitutto evidenziato che l'articolo 13 del decreto-legge reca l'ennesimo intervento per l'ILVA, le cui problematiche si susseguono ormai da anni, rispetto alla quale sarebbe stato forse più ragionevole riflettere e valutare con l'approfondimento necessario tutte le dinamiche connesse all'azienda e rimaste evidentemente irrisolte dai precedenti decreti in materia. Va riaffermato che una disposizione che ripete per la dodicesima volta in cinque anni un intervento per la maggiore industria siderurgica italiana in amministrazione straordinaria, rinnovando deroghe ai codici italiani per consentire la cessione degli *asset* dell'ILVA, rappresenta certamente un modo di operare ancora una volta ai limiti della costituzionalità. L'articolo 14, invece, reca la proroga dei termini previsti dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti. Si unisce questo elemento per evidenziare che il decreto-legge ripropone una serie di disposizioni che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano una evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dal citato articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Approfittando di questo autentico "treno merci varie", quale è lo strumento del decreto-legge, ci si carica sopra di tutto, persino l'articolo 15 che reca disposizioni di carattere meramente organizzativo degli uffici pubblici che non necessitavano di un provvedimento *ex* articolo 77 della Costituzione

che in ogni caso non introduce disposizioni in grado di portare efficacemente, alle Regioni del Mezzogiorno, benefici di natura economica, bensì disposizioni che avrebbero potuto essere applicate in qualsiasi Regione italiana, anche del Nord e anche in Regioni virtuose.

di configurare, mediante una legge di conversione, nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge, nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali. Ora, io mi sono distratto perché non posso seguire tutto: sapevo che erano in discussione norme per lo sviluppo economico del Mezzogiorno d'Italia e con grande sorpresa mi sono trovato una norma adesso sto parlando del metodo ma poi, Presidente, verrò al merito visto che è presente il Ministro degli interni - che considero demenziale. Siamo un Paese dove, se c'è un incidente stradale, si corre a fare una legge sugli incidenti stradali totalmente sbagliata, come è emerso

non erano d'accordo con la sua relazione, si è semplicemente segnalato alla Commissione affari costituzionali che il decreto-legge al nostro esame, così come modificato, è totalmente illegittimo.

Allora, scusate, proviamo a ragionare: come è stato detto anche in Commissione, al contadino che brucia le stoppie - dolosamente, perché non potrebbe farlo - sul suo podere o sul suo fondo, oltre alla condanna, viene anche confiscato il podere,

che questa norma verrà cancellata. Siamo qui per fare le leggi o per leggere il giornale al mattino, vedere qual è la notizia che fa più effetto e correre a fare una norma penale, mai meditata da nessuno, mai vagliata da nessuno, in un pomeriggio, in mezz'ora, tra la Commissione giustizia e la Commissione bilancio? Ma la Commissione bilancio - mi rivolgo al Presidente bilancio? Ma la Commissione bilancio - mi rivolgo al Presidente - è deputata ai giudizi di costituzionalità, nel momento in cui, in un decreto-legge come questo, vengono inserite norme penali, contravvenendo alle disposizioni della Corte costituzionale? E come mai la Commissione affari costituzionali non è stata minimamente interessata all'approfondimento di questo tema? Mi sembra di capire infatti che, essendo già l'emendamento e la sanzione penale introdotti nel testo, se il Governo metterà la fiducia, passerà questo obbrobrio.

perché a questo punto, per correre dietro ai titoli dei giornali, ho l'impressione che questo Senato e questa Camera siano disponibili ad approvare le cose più incredibili. Si tratta però sempre di norme penali e di condanne, con norme sempre più

come si farà a stabilire quando il contratto è stato stipulato correttamente e quando invece c'è un incapace, che in qualche modo è stato imbrogliato, fuori dalla fattispecie della truffa.

Lo ripeto: chi andrà a valutare le responsabilità rispetto a chi sicuramente va a far scoppiare gli incendi lontano da casa sua o dal suo podere, magari per dare la colpa ad altri?

concreta, con tutti gli effetti che può avere, ad un'emergenza occupazionale ed economica nel Meridione, e alla fine far deragliare tutto a causa di una norma di questo tipo, che non è stata vagliata e approfondita da nessuno. Lo so che poi ci sono logiche

cercando di far credere che i problemi vengano risolti sempre con le manette, con la repressione e inserendo nuovi reati. E magari fossero efficaci! Mentre la norma è scritta in maniera tale che qualche poveraccio,

per fare regali e per i saldi di fine stagione!

Dicevo quindi che, siamo di fronte al solito assalto alla diligenza a fini elettorali. Vediamo un po' anche in quelli che sono gli ambiti di mia competenza cosa è successo. Ad esempio, abbiamo visto sbucare un emendamento, che prevede lo stanziamento per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di 4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250.000 euro, a regime, dal 2018 in poi. Ora ascoltate dove sono state prese le coperture per questa misura straordinaria volta a coprire le risorse necessarie per pagare gli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento: sono state prese dal Fondo unico per lo spettacolo dal vivo. Evviva! Quello è il pozzo senza fine, evidentemente, perché da si va sempre a prendere, come se in Commissione non avessimo appena licenziato un provvedimento che prevede addirittura un rafforzamento di quel Fondo. Ma poi, alla fine, quale sarà il risultato di questo rafforzamento se noi continuiamo ad attingere a piene mani da quel Fondo?

Evviva! Già nella buona scuola era prevista tutta una serie di misure a costo zero, ora andiamo a prendere, dalle risorse destinate, altri soldi per il contributo speciale all'Accademia nazionale di Santa Cecilia e un giorno scopriremo a chi stiamo facendo il favore. Tra Tra l'altro, fa ridere tantissimo la motivazione data dalla ex sottosegretaria Vicari per l'inserimento di questa misura all'interno del decreto-legge per il Mezzogiorno, che ha detto che tanti insegnanti dei corsi di perfezionamento all'Accademia di Santa Cecilia sono maestri di musica del Sud e che, quindi, c'è una certa pertinenza con il decreto Mezzogiorno. Poi abbiamo le risorse destinate alle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci. Nutro grande rispetto nei confronti di un gigante simpatico, so che ha organizzato una bellissima mostra fotografica, a Milano, sulla figura di Antonio Gramsci: allora che le iniziative che questi soldi andranno a finanziare siano anche ulteriori, rispetto a quelle organizzate giustamente e - mi dicono - anche con grande competenza dal senatore Ugo Sposetti. abbiamo l'emendamento del Governo 15.0.1000, un aggiuntivo all'articolo 15, che prevede un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a favore delle Province

sarà presa dalle somme impegnate e non più dovute per la carta diciottenni, la famosa 18App. Qui mi scappa da ridere perché, qualche giorno fa, il nostro ex *Premier*,

che è venuta a dirci come stesse funzionando e che erano già stati spesi tanti soldi e che, però, tanti ne rimanevano e che, perciò, stavano valutando l'ipotesi di prorogare questa magnifica iniziativa. E, Oplà: i soldi rimasti dall'iniziativa della carta cultura per i diciottenni vanno a finanziare le Province. Benissimo. È tutto magnifico. Poi abbiamo l'articolo 12, che vuole recepire una sentenza della Corte costituzionale in merito al costo *standard* per studente per il riparto del Fondo per il funzionamento ordinario delle università e, anche qui, si è persa l'occasione

è poi il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa minorile. Certamente è un obiettivo lodevole ed encomiabile, peccato però che non vi siate preoccupati e non abbiate voluto prendere in considerazione dei nostri emendamenti che chiedevano, proprio per raggiungere questo obiettivo, di mappare le tante ricchezze presenti nel Sud d'Italia e di mantenere fede a degli indirizzi dati dalla 7a Commissione, che ha approvato all'unanimità una risoluzione

affinché diventassero centri di aggregazione culturale e di promozione sociale per recuperare quel patrimonio intellettuale ricchissimo di cui il Sud si può fregiare, perché ha tanti giovani bravi che meritano opportunità e luoghi in cui aggregarsi e mettere a disposizione della collettività le proprie intelligenze vivaci.

e ve ne siete fregati di queste proposte che andavano proprio nella direzione di voler integrare questa battaglia e farla diventare a tutto tondo.

per l'anno scolastico 2017-2018 nelle scuole del cratere colpito dal sisma sarà possibile formare delle classi con un numero di studenti minimo in deroga alla normativa vigente, sarà grazie al Movimento 5 Stelle che ha presentato un emendamento a prorogare una deroga contenuta in un provvedimento del gennaio 2017 che si preoccupava giustamente del completamento dell'anno scolastico. Concludo con questa bella notizia che rende tutti noi molto orgogliosi.

colleghi senatori, rappresentanti del Governo, credo che l'importanza di questo decreto-legge meriti un'attenzione, da parte di tutti noi, superiore a quella dimostrata finora,

siano positive solo alcune delle cose che magari si è contribuito ad approvare, grazie a una maggioranza che le vuole e le approva. Il decreto-legge infatti prevede misure allargate, che vanno a incontrare una contraddizione di questo nostro Paese, che ha dimenticato nel dibattito politico e istituzionale la questione meridionale, ma che invece se la ritrova ogni giorno davanti nel suo lavoro costante. Diventa difficile nel dibattito di oggi in Aula, ben introdotto dai relatori, relatori, citare Giustino Fortunato o Salvemini, Saverio Nitti o Antonio Gramsci. Mi limito solo a citare Pertini, nel 1982 messaggio di fine anno), quando sostenne che il problema del Mezzogiorno non può essere considerato solo un problema di quelle Regioni, ma deve essere considerato invece un problema nazionale, se lo si vuole superare. Aveva ragione e ha ancora ragione chi sostiene quelle tesi, differentemente da chi sostiene invece che il Sud sia magari una zavorra per il Paese. Io non lo penso, molti di noi non lo pensano e non lo pensa questo Governo. Tanto non lo pensa, che al suo interno ha un Ministro, dopo anni, che si occupa con competenza di Mezzogiorno non si dimentica che c'è una questione meridionale, perché in questo decreto-legge la affronta in maniera nuova e moderna, non attraverso politiche di assistenza, ma attraverso sostegni per incentivare lo sviluppo dei settori produttivi trainanti e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, necessari l'uno e l'altro a una visione nuova del Mezzogiorno, perché purtroppo le politiche che abbiamo alle spalle hanno solo diminuito alcuni dei divari che ci sono tra Nord e Sud. l'Abruzzo è una Regione che era uscita dal Mezzogiorno, che era uscita dalle contribuzioni europee per il Sud, che ha avuto per un breve periodo una una sorta di uscita morbida, ma che poi è dovuta rientrare, proprio perché le politiche non furono quelle giuste. Oggi l'approccio è nuovo, oggi ci sono misure a favore dei giovani imprenditori, oggi si dà un messaggio chiaro ai ragazzi e si dice loro di restare al Sud, si individuano strumenti e meccanismi, si individuano fasce di età, controlli, tutoraggi, monitoraggi, si individuano i soggetti gestori, si individuano le filiere, si inserisce l'agricoltura all'interno delle possibilità per un giovane di scegliere di rimanere al Sud. Ci sono poi le Zone economiche speciali (ZES), con i porti, che sono dei punti di modernizzazione assolutamente importanti e necessari. Con questo decreto-legge ci siamo esercitati in un lavoro importante in Commissione. Oggi chi si smarca contraddice il comportamento avuto il lavoro costante e quotidiano di queste giornate. Ed è proprio in Commissione che, grazie a una stretta collaborazione con i relatori e con il Governo, abbiamo tirato fuori ulteriori e positive iniziative, che però non vanno a contraddire quelle che già il Governo aveva messo in campo, ma le vanno a precisare e a rafforzare, semmai a dettagliare e a migliorare. Ci sono misure importanti. Vi sono intanto le iniziative per rispondere alle molteplici esigenze delle popolazioni colpite dal sisma 2016‑2017. Sono passati diversi emendamenti; i relatori hanno preso atto di alcune esigenze e le hanno sistematizzate in un emendamento che produce alcune importanti proroghe: la proroga dello stato di emergenza; la proroga per la presentazione dei progetti per gli indennizzi; la proroga per il sistema di recupero e di intervento sui rifiuti e le macerie, con l'aggiunta di nuove risorse pari a 100 milioni di euro. Si approva altresì un emendamento - da me presentato

Alcune norme e alcuni incentivi prevedono risposte forti e certe, certamente migliori e molto superiori a quelle date in altre vicende analoghe. analoghe. Forse dobbiamo rivedere e aggiornare le *governance*, molto complesse e molto irrigidite e che spesso fanno sì che i buoni provvedimenti che approviamo arrivino in ritardo alle popolazioni e ai cittadini.

che non si possa assolutamente rinviare la trattazione delle questioni legate all'emergenza del terremoto, ancora così vicino a noi e ancora così drammaticamente percepito dalla popolazione. Importante - voglio sottolinearlo - è anche un emendamento presentato dal Governo, recependo azioni importanti provenienti dalla Regione Abruzzo e dalla mia modesta attività parlamentare, che stanzia 250 milioni per la sicurezza delle autostrade A24 e A25. Mi voglio soffermare su questo provvedimento, perché quelle autostrade che collegano l'Abruzzo al Lazio, fortemente trafficate a causa di un quotidiano movimento di migliaia e migliaia di persone che si muovono dall'Abruzzo al Lazio e viceversa,

non solo danni al territorio, ma anche, purtroppo, a quelle autostrade. La sicurezza va garantita e questo provvedimento del Governo va incontro ad esigenze più volte richiamate, ma saranno sicuramente necessari ulteriori provvedimenti. In tal senso ho presentato un ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo, perché si prenda atto di una situazione particolarmente delicata e di emergenza, anche alla luce di una sentenza del TAR, intervenuta proprio oggi, che sconfessa l'azione del Governo e autorizza Autostrada dei parchi a poter aumentare i pedaggi. Questo potrebbe produrre sui cittadini che quotidianamente percorrono su questi assi autostradali un ulteriore incremento delle tariffe, che dobbiamo assolutamente scongiurare. Le misure contenute in questo decreto-legge, quindi, spaziano su più possibilità e su diverse aree di intervento economico. Intervengono anche sulla dispersione scolastica e su problematiche gravi, da decenni, che riguardano il Mezzogiorno d'Italia, la crisi economica, in particolare di determinate aree, e la crisi sociale spesso connessa alla crisi economica, che porta molti ragazzi a un abbandono precoce del sistema scolastico e comunque alla condanna, purtroppo per loro stessi, a dovere fare i conti con un sistema sociale senza nemmeno i titoli di studio di base. Anche da questo punto di vista nel decreto-legge ci sono misure importanti, rafforzate dall'intervento emendativo di colleghi del Gruppo Partito Democratico, che voglio sottolineare per la loro sensibilità e per la loro importanza. Oltre a questo, venivano giustamente richiamati gli altri strumenti che abbiamo messo in campo, Governo e Parlamento, per il Sud,

dalle istituzioni, spesso in stretta collaborazione tra di loro, possano poi avere un dispiegamento, un esercizio di concretezza nei territori in tempi più rapidi e più adeguati alla necessità di quegli stessi territori, dove non si fugge più con la valigia di cartone legata dai lacci, ma dove si fugge - ancora, purtroppo - spesso con il *computer*, con i titoli di studio, con i *master*, alla ricerca di altri spazi e di altre possibilità. Ecco, però, che per rispondere proprio a queste nuove esigenze, a queste nuove drammatiche fughe, non si possono adottare strumenti vecchi, assistenziali,

all'opposto di vecchie pratiche clientelari e assistenziali, ad incidere proprio nelle aree problematiche (ma che vengono individuate come aree di potenzialità di sviluppo) a mio avviso

la verifica degli strumenti adottati e con i necessari aggiustamenti, se dovessero servire. Nello studiare le misure adottate

proprio per evitare che lo sforzo titanico che questo Paese sta facendo per dare risposte a quelle popolazioni non venga poi annullato

per dare ulteriori spazi, certezze, fiducia e futuro a quelle popolazioni. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge giunto all'esame dell'Assemblea segue quello dello scorso dicembre, con cui il Governo ha avviato una campagna di aiuti per le situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. in esame si è resa necessaria per la necessità di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle Regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, introducendo misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione. Per quanto riguarda le misure di incentivazione all'imprenditoria giovanile, significativa è la misura «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Si prevede un finanziamento fino a 1.250 milioni di euro per i nuovi giovani imprenditori *under* 35 del Sud Italia e di 50 milioni di euro per favorire gli imprenditori agricoli *under* 40. Sono inoltre previsti circa 200 milioni di euro per le Zone economiche speciali (ZES), 40 milioni di euro per favorire le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e 150 milioni di euro per il sostegno amministrativo agli enti locali. Queste azioni, come capisaldi del provvedimento di urgenza, hanno l'obiettivo di dare un maggiore impulso all'economia del Mezzogiorno, alla cultura imprenditoriale e all'innovazione delle Regioni del Sud, in linea con il processo già avviato con il precedente decreto-legge promuovere l'individuazione di nuovi incentivi per i nuovi giovani imprenditori e l'introduzione di procedure semplificate. Con la misura «Resto al Sud» ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, di cui il 35 per cento come contributo a fondo perduto, erogato dal gestore della misura, e il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, rimborsato entro otto anni dalla concessione del finanziamento. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative alla produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero alla fornitura di servizi, ivi compresi quelli turistici. inoltre previste azioni di accompagnamento da parte di enti pubblici, università e associazioni del terzo settore a supporto di questo processo di crescita. Chi sarà in grado di produrre progetti credibili e sostenibili, avrà il pieno appoggio dello Stato, in un rapporto di responsabilità reciproca. Con il presente decreto-legge si cerca inoltre di rivalorizzare terreni abbandonati o incolti e immobili in stato di abbandono. Si tratta, in particolare, di terreni agricoli su cui non sia stata esercitata l'attività agricola da almeno dieci anni, di terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree e, infine, di aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, nonché delle relative unità immobiliari che risultano in stato di abbandono da almeno quindici anni, o su cui non risultano più operative aziende o società di almeno quindici I Comuni, quindi, devono provvedere a una ricognizione complessiva dei beni immobili e dei terreni agricoli da integrare anche con gli elenchi della Banca delle terre agricole tenuti a livello regionale. I beni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta, ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione dell'utilizzo del bene. sottolineate anche le misure attuate per fronteggiare i danni causati dal coleottero xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi della Regione Siciliana, nonché i danni causati dal batterio xylella fastidiosa per i settori vitivinicolo vitivinicolo e oliario e tutti quelli derivati dalla diffusione nel settore vitivinicolo, tutti settori di estrema rilevanza per il Sud Italia. Per ciò che concerne l'istituzione di Zone economiche speciali, le nuove imprese e quelle già operanti possono beneficiare non solo di semplificazioni di tipo amministrativo, a patto di incrementare gli investimenti oppure di intraprendere programmi imprenditoriali, ma anche del *bonus* Sud, maggiorato rispetto a quello previsto dall'ultima legge di stabilità, per l'acquisto di beni strumentali nuovi che sono destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno. Con il lavoro della Commissione bilancio, a cui va il mio ringraziamento, si è consentita non solo la possibilità di presentare sino a due progetti per Regione relativi alla ZES, ma si è data anche la possibilità alle Regioni del Sud non strettamente collegate con la rete transeuropea TEN-T) di avere una Zona economica speciale interregionale. Per l'esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo e di impresa. In particolare, potranno usufruire di procedure semplificate, dell'accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico della ZES e saranno destinatarie di agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito di imposta al Sud. Infine, è da segnalare anche l'introduzione di strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, nonché la presenza di una misura di sostegno per gli enti locali che accolgono i migranti, in modo tale che nelle situazioni di emergenza questi Comuni non vengano lasciati in balia di sé stessi. Un altro settore essenziale per il Sud e sul quale il provvedimento è intervenuto è la pesca. Con un emendamento approvato in Commissione, sono state finanziate le indennità giornaliere per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivanti da arresti temporanei non obbligatori della stessa. Sul tema ambientale, considerata l'emergenza siccità ed incendi in questi giorni, un ottimo risultato è stato raggiunto con l'inasprimento delle misure restrittive chi incendia terreni a fini ritorsivi. Alternativa Popolare ha visto, con l'emendamento approvato in Commissione, riconosciuta la bontà della questione sollevata durante la fase emergenziale, dando una risposta concreta ad una piaga che sta affliggendo le nostre aree boschive. Per concludere, signora Presidente, vorrei sottolineare una delle tante risposte che l'Italia ha dato sul tema della sicurezza nei centri delle città. Nel presente decreto-legge abbiamo previsto un controllo in entrata ed in uscita dai centri storici delle Città metropolitane dei flussi di merci mediante la realizzazione di un sistema automatico di controllo che sfrutti un nuovo modulo della piattaforma logistica nazionale. Questo è uno strumento per conciliare, al contempo, sicurezza e turismo. I flussi turistici, pertanto, non saranno compressi, ma la loro permanenza ed il loro fluire saranno garantiti da un ulteriore strumento all'avanguardia. In merito al Sud Italia, penso immediatamente ai casi di Palermo, in qualità di capitale della cultura italiana 2018, e di Matera, in qualità di capitale della cultura europea 2019. Questo provvedimento, tanto atteso dalle Regioni meridionali, si pone ormai in un processo costante di valorizzazione delle eccellenze e dei punti di forza del Meridione e di stimolazione delle forze e delle capacità dormienti del nostro Paese. Pertanto, non posso che auspicare una rapida approvazione del provvedimento.

veramente noi ci chiediamo quale sia l'interesse del Governo, della maggioranza e dello stesso Parlamento per la cosiddetta questione meridionale, che è una questione nazionale. Questo è un provvedimento Dal momento che andiamo a destinare 20 miliardi di euro per il risanamento delle banche del Nord, delle banche venete, del Monte dei Paschi, delle banche del Centro-Nord

non esiste una possibilità di attenzione. Nessuno chiede assistenzialismo, ma non c'è una strategia. Non c'è una direzione; non esiste una valorizzazione delle grandi potenzialità del del Mezzogiorno nel panorama complessivo europeo e mediterraneo. Nessuno parla dei grandi traffici internazionali, nessuno parla del

Siamo tornati ai vecchi concetti postbellici dell'occupazione delle terre, attraverso l'intervento sulle terre incolte. Non ci si chiede, però, perché esistano ancora, nel nostro Paese, terre

dell'economia nazionale e dove ancora migliaia e migliaia di ettari vengono annualmente sottratti all'attività agricola dall'espansione urbanistica, perché esistano ancora terre incolte. Ma esistono? O questo è uno strumento, di stampo molto caro alla sinistra, per camuffare un'azione espropriativa soprattutto sugli immobili? Le terre, infatti, hanno talmente poco valore che ben poco possono produrre in termini economici a chi, eventualmente, va ad utilizzarle, ove mai questi progetti e queste situazioni si possano concretizzare. Vi sono, però, immobili che sappiamo essere oggetto di occupazione abusiva già da ora, soprattutto in alcune grandi città; e sappiamo benissimo da chi e per quali fini sono occupate. Questo è un cavallo di Troia per legalizzare situazioni assolutamente illegali? Ma, a parte questo, conoscenza, anche attraverso la lettura del resoconto dei lavori della Commissione, di tutta una serie di interventi che con il Mezzogiorno non hanno nulla a che vedere peggio ancora, con esso hanno a che vedere e sono risolti nella maniera sbagliata, non incidendo cioè sulle cause ma andando, come sempre, a cercare di imporre situazioni, soprattutto di carattere penale, penale, che abbiamo dimostrato non essere risolutive di quelli che sono i mali. Ancora una volta si verificano gli incendi? Bene, cosa pensano di fare la maggioranza e il Governo?

all'abolizione del Corpo forestale dello Stato, voluta come capriccio semplificativo, che poi tale non è stato, da parte del precedente Governo e da parte di questa maggioranza perché bisognava dare un segnale

cari colleghi, lo ripeto, se questa è la politica del Governo per il Mezzogiorno, aliena da qualsiasi intervento strutturale, aliena da qualsiasi intervento strategico, aliena dal vero interesse delle popolazioni del Mezzogiorno,

uno scatto d'orgoglio. Come si suol dire, si fa di necessità virtù, e quindi l'abbandono, in questo caso, può fare virtù. Noi confidiamo sempre nel fatto che le popolazioni del Mezzogiorno abbiano un loro scatto di orgoglio. In questo caso non può che essere uno scatto che parte dalla

Paese. Se questi sono veramente i provvedimenti per il Mezzogiorno, allora bisogna chiudere questo decreto-legge. Lo voterete voi con il voto di fiducia (ma non certamente con la fiducia delle popolazioni del Sud). Mi chiedo se, nell'ambito della maggioranza, i colleghi che vengono dal Mezzogiorno d'Italia dicano

Questo è purtroppo ciò che ha condannato il Sud dall'unità d'Italia fino ad oggi. Noi stessi siamo stati artefici della nostra arretratezza perché abbiamo subordinato

scelte che privilegiassero, soprattutto in termini infrastrutturali, altre zone del Paese. Quindi, fino a quando continueremo a rimanere, come classe politica del Sud, ingabbiati in questa in questa cintura, in questa camicia di forza costituita dall'obbligo del rispetto delle maggioranze e dall'obbligo del rispetto delle direttive che vengono dalle segreterie politiche che che costringono coloro che fanno parte della maggioranza ad accantonare gli interessi del Mezzogiorno pur di privilegiare gli interessi politici generali, sicuramente il Mezzogiorno non avrà alcuna

finanziare la decontribuzione sulle nuove assunzioni, che poi ha creato una bolla occupazionale della quale pagheremo, alla scadenza del provvedimento, sicuramente gli effetti a livello complessivo nazionale, sono stati bloccati 4 miliardi e mezzo di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno nell'assoluto silenzio

con gli occhi bassi i miei colleghi, sia della mia Regione che di altre Regioni meridionali, votarono a favore del provvedimento proposto dal Governo dal Governo di centrosinistra dell'epoca. Questo sarebbe bastato a restituire al Mezzogiorno il maltolto di una rapina

e non avranno prodotto alcuna reale modifica della situazione economica del Mezzogiorno. Fino a quando ci accontenteremo, per così dire, di tutto questo e vedremo passare

l'obiettivo di questo provvedimento è dare maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nei territori del Mezzogiorno. Tale progresso non può prescindere dallo sviluppo educativo, tema trattato in alcuni articoli a cui mi riferirò in modo specifico. L'articolo 11 consente al MIUR di individuare, a seguito di un decreto e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, giustizia, aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata, per poter poter emanare dei bandi che saranno rivolti a reti di scuole in convenzione con gli enti locali, soggetti del terzo settore, strutture sportive territoriali, o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Lo scopo è quello di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi di durata biennale in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Ce lo dicono anche i dati riportati dal IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017, che mostrano come in Italia la condizione di persone di minore età che vivono in condizioni di povertà assoluta sia peggiorato. Il peggioramento diffuso delle condizioni economiche ha colpito le persone più vulnerabili e tra questi i minori e le nuove generazioni che hanno pagato il prezzo più alto. I dati a nostra disposizione fanno emergere quanto i rischi e le fragilità siano reali e, di conseguenza, quanto gli interventi atti a combattere i fenomeni presi in esame dall'articolo 11 del provvedimento in discussione siano prioritari quanto urgenti. Non possiamo creare sviluppo se non partiamo dall'educazione, dalla cultura e dalla conoscenza. E sappiamo che la povertà minorile non riguarda solo il Sud e non riguarda solo l'educazione. Sono temi che trattiamo da anni in Commissione istruzione e cultura e nella bicamerale infanzia e adolescenza, con indagini conoscitive sia sulla povertà che sui diritti al patrimonio culturale ed artistico. Sono temi che abbiamo affrontato con provvedimenti importanti del Governo che riguardano sia la scuola, sia gli affari sociali: pensiamo, per esempio, ai bandi per la povertà educativa che sono stati emanati quest'anno e porteranno risorse laddove ci sarà bisogno di lavorare in questo senso. Il rischio per i minori è associato in primo luogo alla ripartizione geografica di residenza e al titolo di studio della persona adulta di riferimento, come riporta la relazione al Parlamento di quest'anno del Garante dell'infanzia dell'adolescenza. Quindi, conta dove vive un bambino e che titolo di studio hanno i suoi genitori. hanno i suoi genitori. I minori nel Mezzogiorno e quelli che vivono in famiglie con a capo una persona che ha al massimo la licenza elementare presentano infatti un rischio di povertà relativa di circa 4 volte superiore a quello, rispettivamente, dei residenti nel Nord e di quelli che vivono con una persona di riferimento almeno diplomata. Sempre dal rapporto apprendiamo che, in conseguenza al maggiore impatto dei flussi migratori nelle Regioni meridionali, oltre il 60 per cento dei minori non accompagnati trovano accoglienza nelle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata: anche a questo devono fare fronte pubblicato da Save the Children nel 2017, che è già stato menzionato, si desumono alcuni dati rispetto ai ragazzi di quindici anni, che non raggiungono le competenze minime in matematica e in lettura. Si evince che un adolescente che vive in Campania ha quasi il doppio di probabilità di non raggiungere le competenze minime in matematica rispetto ad un coetaneo che vive in Lombardia il triplo rispetto ad un quattordicenne delle Province autonome di Bolzano e Trento. Percentuali molto simili si riscontrano riguardo alla lettura:

riconosciuto dai progetti europei come buona pratica, grazie al quale il tasso di dispersione scolastica si è abbassato di due punti percentuali in cinque anni. È possibile intervenire ed avere risultati concreti, ma è necessario costruire sistemi di rete con gli enti locali, il privato sociale e gli enti culturali, come indica l'articolo 11 del decreto-legge Oltre alle condizioni di povertà assoluta e relativa, sempre nel rapporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono emersi segnali allarmanti per i casi di povertà educativa, in riferimento non solo al sistema di istruzione formale ed informale, ma anche rispetto al diritto alla crescita e allo sviluppo relazionale, affettivo ed emozionale. Ecco perché è più opportuno parlare di povertà educative. Nel nostro un minore su 10, tra i sei e i diciassette anni, nel 2016 non è mai andato al teatro o ad un museo, non ha mai visitato mostre, monumenti e siti archeologici, non ha fatto sport con assiduità. Sono sei su 10 coloro che non hanno svolto quattro o più delle attività menzionate e i picchi sono in Calabria, in Sicilia e in Campania. Quindi il decreto-legge al nostro esame entra proprio in questo merito.

coerente con il livello di efficienza dei costi sostenuti dagli atenei per erogare i propri servizi agli studenti. I lavori della Commissione in

del Mezzogiorno. In particolare, ricordo l'emendamento sulla dotazione *standard* della docenza, che la determina in modo che la stessa rimanga "costante" nell'ambito di un certo *range* di numerosità degli studenti per ogni classe di corso di studio. È stato precisato che i diversi contesti ai quali riferirsi per la valutazione della diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, con riguardo al reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo, di norma a livello regionale, siano in particolare quelli «economici e territoriali». Ancora, è stato previsto che il costo *standard* per studente di ateneo sia moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio, cui si aggiungono, come è già stato detto in quest'Aula, anche gli studenti iscritti al primo anno fuori corso. Desidero ulteriormente focalizzare due punti e concludo. Il primo riguarda i *cluster* tecnologici nazionali. È stato approvato in Commissione un emendamento importante, che si occupa dei *cluster* tecnologici nazionali, quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. Si tratta di figure riconducibili a poli di innovazione di cui al Regolamento UE della Commissione, dovranno presto assumere la forma di associazione riconosciuta o fondazione, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro. È previsto che ciascun *cluster* elabori un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descriva le attività che che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre

per poter dare continuità alla deroga rispetto all'organico degli insegnanti anche per l'anno scolastico 2017-2018.

Questo va detto perché colloca così in modo opportuno il provvedimento che, ripeto, giudico positivamente per ciò che può fare nelle condizioni date. Non è un provvedimento che esaurisce un percorso necessario; è un provvedimento che accenna ad alcune questioni che vanno trattate in maniera più coordinata e omogenea in una politica per il Mezzogiorno di cui noi abbiamo bisogno e che non possiamo più tardare a mettere in campo.

riferisco all'intervento sull'occupazione giovanile, sull'autoimpiego e sull'autoimprenditiorialità

utilizzando le forme di finanziamento possibile, sia quelle a fondo perduto sia con il credito a tasso d'interesse agevolato, anzi addirittura totalmente abbattuto. inoltre, partendo dalla convinzione che bisogna valorizzare lo sviluppo locale, cioè le vocazioni produttive dei luoghi, le risorse che sono distribuite in un'area del Paese che rimane povera, ma che è ricca di potenzialità, di qualità. Questo se noi la difendiamo.

il patrimonio di tutti, ricondurre la terra alla sua originaria funzione, cioè quella della produzione, che la vuol salvaguardare dagli inquinamenti. C'è chi difende il territorio, ma c'è anche chi lo aggredisce, chi agisce sulla spinta degli egoismi personali e sulla base delle ambizioni irrefrenabili verso la ricchezza, verso l'accumulazione, verso un uso proprietario del bene comune. C'è chi ha questo approccio e chi invece difende il patrimonio comune. Io credo che su questa linea favorire l'autoimprenditorialità, anche in settori delicati come l'agricoltura,

fossimo all'interno di quella logica, perché c'era il senso di essere popolo, di essere impegnati ad affrancarsi dalla povertà e a ricostruire un Paese dilaniato dalla guerra civile e dai lutti della Seconda guerra mondiale. Io penso che quella sia stata una stagione assolutamente produttiva di cui dobbiamo tenere memoria a 360 gradi, riconoscendo le cause delle difficoltà di quell'epoca, ma anche i meriti in quella situazione della voglia di riscatto che si è registrata in Italia e di voglia di riscatto noi dobbiamo parlare per il Mezzogiorno quando affrontiamo questo tema. Lo sviluppo locale è una grande cosa, perché mette nelle mani di chi vive nei luoghi la possibilità di organizzare la propria esistenza. Del resto, l'occupazione che noi evochiamo non la possiamo più ritrovare

Partire dallo sviluppo locale, cioè costruire le condizioni di sviluppo dove si vive e ancorare l'attività economica al destino del proprio territorio, significa partecipare alla vita della comunità costruendo, per quella comunità, una prospettiva di progresso. Questo è quello che in parte c'è in questo provvedimento, che ha ancora il carattere di emergenza, che interviene cioè in una situazione molto complicata tentando di inserire qualche elemento positivo, ma sicuramente non decisivo.

Ogni volta che noi facciamo una produzione normativa, ciascuno di noi porta avanti istanze di categorie sociali e di ambiti territoriali, ma si scontra con una realtà abbastanza cruda, di un Governo qualche volta ostaggio anche dei Ministeri. Quando parlo di Ministeri, parlo di quell'insieme di disposizioni e di visioni che sono frutto ormai consolidato dei condizionamenti

la politica, il Parlamento, la capacità di legiferare in funzione del bisogno non possono trovare sistematici ostacoli a concludere cose che servono. Ne cito una per tutte: il Mezzogiorno ha una situazione di infrastrutture e trasporti difficilissima e complicata. Ebbene, signor

anche il sistema delle ferrovie cosiddette complementari, quelle a binario unico, quelle dove si consumano spesso gli incidenti ferroviari più gravi e dove si realizzano i lutti

tale organo, che vale per la dimensione nazionale, valesse anche per le dimensioni regionali e locali del Mezzogiorno d'Italia, dove prevalentemente d'Italia, dove prevalentemente quei soggetti gestiscono il trasporto ferroviario. È una cosa ovvia, che costa un'integrazione di risorse finanziarie a un'agenzia dello Stato.

siccome abbiamo problemi di copertura e abbiamo problemi di riorganizzazione, cosa lasciamo? Lasciamo le ferrovie a gestione locale e regionale fuori dai parametri della sicurezza. Poi, quando si verifica un incidente,

al Ministro di turno di intervenire su una situazione che avremmo potuto regolare, se non avessimo affrontato il problema Lo abbiamo fatto positivamente in un altro caso. La Sardegna è una delle Regioni attraversate dal fuoco

di cura del bosco, di pulizia, di risanamento e di ripristino ambientale dei luoghi. Rischiava di non poterlo fare con costi a carico della Regione e degli enti locali sardi, badate, quindi senza attingere alle casse dello Stato, solo perché esiste una disposizione che impone rigidi limiti alle assunzioni da parte degli enti locali, anche quando si tratta di progetti temporanei, con applicazione temporanea di personale e del tutto occasionale. In questo caso ci si è venuti incontro e siamo riusciti ad ottenere la proroga di una disposizione che avevamo già messo in campo in in circostanze anche allora difficili, quelle dell'alluvione di Olbia e dei lutti che da esso sono venuti, proprio perché c'era un problema di cura e manutenzione del territorio.

facendo una manutenzione accurata di quel territorio e salvaguardandolo dalle possibili aggressioni speculative.

Va fatta notare una prassi di questa maggioranza,più attenta alla ricerca di titoli roboanti che di contenuti finalizzati a cambiare realmente le cose. Così, mentre le banche negli ultimi anni hanno incassato ben 85 miliardi di contributi a fondo perduto dallo Stato, per il rilancio di mezza parte del Paese quanto avete stanziato? Poco più di 1 miliardo, di cui la maggior parte viene dai fondi per lo sviluppo e la coesione indicati nella legge di stabilità 2014. Finalmente avete speso questi soldi, che sono pochi e spesi male. Come si fa seriamente a favoleggiare la ripresa del Sud praticamente con le briciole, di quello che rimane dopo una serie di provvedimenti che non fanno altro che trasferire ricchezza dai cittadini italiani a poche grandi imprese? Giusto per capire quali sono le priorità di questo Governo e di quelli che l'hanno preceduto, ovvero le banche, va detto che tra i giovani e meno giovani del Sud e le banche, avete scelto queste ultime. Altro che discorsi pomposi, che dai noi in Sicilia si definiscono discorsi da «quaquaraquà», per citare il famoso Sciascia, che tutti noi ben conosciamo. Quindi tanta retorica ma pochi fatti, come piace al PD. Il Sud è pieno di emergenze, ma voi lanciate la misura «Resto al Sud», che dovrebbe incentivare i nostri giovani a rimanere al Sud, ad aprire piccole e medie imprese. Davvero, io sono convinta che molti di voi abbiano sbagliato mestiere: dovevate tradurre i titoli dei film esteri; altro che lavorare in questo Palazzo! «Resto al Sud», ricorda molto «Benvenuti al Sud», una fortunata pellicola, comica quanto questo decreto-legge. Uno degli ingredienti sono i giovani, quelli con le tre G davanti, che rendono benevola ogni iniziativa. Chi se ne frega se uno dei problemi del Sud sono i meno giovani, altrettanto bisognosi di incentivi? E giù di retorica inutile e controproducente. Noi, che siamo responsabili, abbiamo proposto una serie di modifiche, a partire dalle condizioni basilari per rimanere al Sud: avere un'abitazione dignitosa. Ho presentato un emendamento che chiede di recepire un mio disegno di legge che riguarda l'autorecupero di immobili abbandonati sia pubblici che privati, per recuperare i centri storici delle nostre città di Provincia abbandonate, magari instaurando attività artigianali e inserendoli in percorsi turistici. questo emendamento richiede una spesa poco superiore ai 400 milioni di euro che non prenderemo dalla fiscalità generale, bensì da piccoli aumenti delle aliquote a banche e assicurazioni, che sono le uniche entità che in questi anni hanno percepito enormi fondi provenienti dallo Stato. Cosa vogliamo fare, signor Presidente, illustri colleghi? Vogliamo recuperare questo patrimonio edilizio e dare in comodato d'uso una casa a chi ne ha bisogno o vogliamo che i nostri giovani, che già sono senza lavoro, non abbiano nemmeno una casa, cosi sono super incentivati ad andare via? Ha ragione chi ha presentato pregiudiziali di costituzionalità: in questo decreto-legge avete messo di tutto, finanche i soldi per la solita emergenza migranti. Anche in questo caso, però, avete sbagliato, a mio modesto avviso, perché, invece di dare soldi e incentivare i Comuni che accolgono, avete semplicemente aumentato i fondi per l'accoglienza, creando ulteriore disparità tra i cittadini italiani, a cui continuate a negare il reddito di cittadinanza e il lavoro, e gli amici degli amici che li accolgono, che avranno ancora più fondi. Nell'emendamento presentato, a mia prima firma, chiedo invece di togliere i vincoli alle somme destinate ai Comuni per devolverle a quei Comuni che accolgono come fondi da spendere per i propri cittadini non per l'accoglienza; ma anche in questo caso mi pare che non ci siamo.

a quindici anni, equiparando di fatto l'incendio boschivo al terrorismo; bisognava aumentare i vincoli per i terreni bruciati al punto da rendere antieconomico appiccare il fuoco, e invece avete introdotto una norma liberticida che sequestra il terreno all'agricoltore per darlo al Comune che non sa assolutamente cosa farsene. Complimenti vivissimi! *(Applausi

necessarie a stimolare la crescita economica del Mezzogiorno. Ebbene, l'urgenza è una condizione stabile nel nostro Mezzogiorno, dai tempi dell'Unità d'Italia. Protagonista è oggi, ancora una volta, la questione meridionale, e cioè l'insieme dei problemi posti dall'esistenza del Mezzogiorno, ma vi anticipo sin dall'inizio del mio intervento che la questione è ben più ampia e non riguarda il solo polo Sud dell'Italia. Sud dell'Italia. Oggi c'è una situazione per cui si registra un più basso livello di sviluppo economico, un diverso e più arretrato sistema di relazioni sociali, un più debole svolgimento di molti importanti aspetti della vita civile rispetto alle altre Regioni del Paese, in particolare quelle settentrionali. Il grave degrado della vita amministrativa e i sistemi di poteri locali, l'indigenza in cui versano nel Mezzogiorno i nostri concittadini rappresentano uno dei più gravi fallimenti dello Stato, frustrate le ricette proposte dalla destra storica, dalla sinistra trasformista, dal giolittismo, dal fascismo, dal compromesso storico fatto di cassa del Mezzogiorno, finanziamenti a pioggia, cattedrali nel deserto, consenso clientelare, autarchia particolaristica che ha allontanato gli investimenti privati senza portare a profitto gli ingenti investimenti pubblici. C'è oggi bisogno di misure che riducano il differenziale di crescita delle zone più depresse del nostro Paese, di tutte le zone del nostro Paese ovunque siano collocate geograficamente. Occorre andare oltre gli stretti confini geografici. Per realizzare questo obiettivo sono necessarie riforme di struttura che intervengano e invertano radicalmente la tendenza in corso in tutto il Paese, non solo al Sud. C'è poi un elemento specifico di critica a questo decreto-legge. Rischiamo di fallire l'obiettivo prefissato perché, pure apprezzando lo sforzo economico-finanziario messo in campo dal Governo, mi pare che il provvedimento contenga manovre solo sperimentali, emergenziali, non strutturali, che rischiano di essere insufficienti per dare soluzione stabile al problema annoso. Ciò che facilita la nascita e la crescita di nuova imprenditorialità è sempre utile, ma - lo ripeto - la nuova imprenditorialità sarà concentrata in particolari zone, senza garantire la crescita uniforme dell'intero territorio meridionale, meridionale, né tantomeno sarà utilizzabile nel resto d'Italia. Nel provvedimento è infatti prevista l'istituzione delle Zone economiche speciali sperimentali (ZES), da costituirsi nelle sole aree portuali. Parzialmente utile è anche la misura «Resto al Sud», perché offre ai giovani meridionali che non dispongono di mezzi propri per avviare un'attività produttiva una dotazione di 50.000 euro, un terzo della quale a fondo perduto, e la restante parte concessa con finanziamento a tasso agevolato. Dispiace, però, che si siano voluti premiare il coraggio e l'intraprendenza solo di alcuni dei nostri giovani, ossia dei giovani imprenditori. Mi domando perché siano stati ingiustamente esclusi dai benefici i liberi professionisti e i commercianti, alimentando ulteriori squilibri all'interno del nostro tessuto sociale meridionale. Vengo ora rapidamente al punto che mi appare centrale per criticare la norma che dobbiamo convertire in legge. Mi appare riduttivo e anacronistico concentrare gli sforzi per migliorare la situazione economica dei nostri concittadini proseguendo nell'utilizzo del solo criterio geografico. Sono molti i Meridioni d'Italia e non tutti si trovano al Sud. Mi riferisco alle zone depresse, dove c'è insufficiente attività di impresa perché disincentivata, ostacolata e negata, con le ovvie conseguenti ripercussioni sul lavoro, o, meglio, sulla sua mancanza, ovunque esse si trovino su tutto il territorio nazionale. Ritengo che lo Stato debba intervenire ovunque vi sia bisogno, senza distinzione di latitudine geografica. Un criterio, una bussola per l'intervento pubblico nell'economia potrebbe essere rappresentato dalla media dei dati economici. in tutte le Regioni d'Italia, ovunque il tasso di disoccupazione superi la media nazionale dovrebbero applicarsi misure di favore analoghe a quelle che stiamo per approvare. Faccio l'esempio della mia Regione, le Marche, che ben conosco. Il tasso di disoccupazione più grave e preoccupante negli ultimi anni ha superato la percentuale del 36 per solo la metà degli *over* 50 ha un'occupazione stabile. Più in generale, i dati dell'economia nel suo complesso sono preoccupanti. I dati diffusi dall'ISTAT mostrano una variazione reale del PIL ingravescente negli anni e, quindi, uno stallo dell'economia regionale, in controtendenza rispetto al *trend* nazionale. Si badi bene, i dati non considerano il fatto che il sisma dello scorso anno ha reso drammatica la situazione della Regione, anche se non ancora registrata dall'Istituto nazionale di statistica.

della devastazione ultima del terremoto. Lo stesso valore del PIL procapite marchigiano è inferiore alla media nazionale e pone la Regione e i suoi abitanti in grave difficoltà. Stiamo parlando di una Regione che era ricca. Nel 2008 avevamo tutt'altri parametri. Attualmente le Marche crescono meno della media italiana, solo

viste le esportazioni all'estero. La Regione fatica ad agganciare la ripresa. Ciò ha cause precedenti al devastante sisma che ci ha colpiti, nonostante le Marche siano una Regione vocata alla produzione di eccellenza.

anche se - finalmente - lievissimi segnali di ripresa, grazie all'estrema laboriosità delle genti che la popolano, iniziano a vedersi. Si consideri che le Marche si caratterizzano per l'altissimo tasso di imprenditorialità, potendo vantare un'impresa circa ogni dieci abitanti. Le imprese sono 152.000 e i distretti produttivi sono specializzati nella manifattura di tradizione, dal legno, al mobile al Nord, alla meccanica e agli elettrodomestici, a strumenti di precisione al Centro, nonché al calzaturiero e all'alimentare al Sud. Le imprese un tasso di ricchezza inferiore alla media nazionale, poco inferiore ai 25.000 euro di PIL procapite. La crisi ha ridotto di 20 punti la produzione industriale dal 2008 a oggi, con un tasso di disoccupazione che di più del 10 per cento del complessivo, pari a oltre un terzo degli occupati legati al settore industriale. Si può dire uno *tsunami* sociale, un sisma economico, una devastazione complessiva. Naturalmente, sull'economia regionale ha pesato anche il recente, sciagurato fallimento di Banca Marche, primo istituto di credito del territorio, e di Banca Veneto, aggiungo. Purtroppo, la spesa per ricerca e sviluppo e la quota di imprese *high-tech* - il futuro di qualsiasi Paese voglia rimanere al passo coi tempi - è sotto la media nazionale. Unica nota positiva è rappresentata dalle *start-up* innovative, a dimostrazione che l'*humus* sociale è naturalmente imprenditoriale, se solo si offrissero le condizioni per utilizzare al meglio tutte le potenzialità dei cittadini lavoratori ed imprenditori marchigiani. Per riprendere il percorso di crescita, è necessario un piano strutturato di politica industriale che detti tempi e metodi, interventi e risorse per riprendere un percorso virtuoso di sviluppo in tutte le Regioni d'Italia, non solo nel Mezzogiorno. Ciò vale in particolare anche nelle Marche, per il beneficio della Regione, che può essere propulsore di crescita, favorendo la ripresa di tutto il Paese, attraverso l'emanazione di norme in grado di realizzare programmi basati su meccanismi efficaci di *governance* che coniughino le strategie di programmazione nazionale con le specificità territoriali. Ciò è necessario non tanto e non solo per motivi di miope ed egoistico campanilismo, quanto perché le Marche rischiano lo spopolamento. Il terremoto ha fatto emergere con maggiore forza le debolezza e le criticità territoriali già esistenti nelle aree interne. È chiaro, quindi, che in assenza di una rapida e valida proposta di rilancio, c'è il rischio di un rapido spopolamento, di una delocalizzazione delle attività produttive dalle Marche. Il sisma ha sicuramente accelerato i processi di abbandono del territorio, con relativo degrado del tessuto produttivo e sociale già in atto nelle zone interne. Se tutto ciò si vuole evitare, lo sviluppo futuro di queste aree deve prevedere una programmazione che superi il semplice ripristino dell'esistente, dando efficace soluzione alle problematiche caratteristiche delle aree interne regionali, supportate da una serie di misure specifiche per il rilancio delle attività del territorio. Ne va anche dell'equilibrio idrogeologico dell'Appennino centrale, dell'ecosistema, della tutela della biodiversità, quindi della nostra storia e del nostro futuro, fatto di produzione di eccellenza e - speriamo - di popolazioni stabili e laboriose, capaci di attrarre, grazie alla bellezza del nostro territorio, cittadini stranieri villeggianti, in grado di diventare *testimonial* della nostra eccezionale specificità regionale e nazionale. Onestamente, mi stupisco del fatto che un Governo che ha finto di aver capito le reali necessità del nostro Paese, cioè il Sud dell'Europa, che ha lasciato credere di aver compreso il bisogno della società e dei cittadini si affrontassero seri interventi di sostegno strutturale dell'economia reale, invece, quando poi ha avuto la possibilità di emanare un serio ed efficace provvedimento a sostegno del Sud e dei suoi abitanti, non abbia voluto seriamente analizzare la realtà per dare una soluzione, negandosi così la possibilità di affrontare e risolvere le reali problematiche Questo Governo si è limitato ad autodelegarsi, per rifare gli errori del passato, per riproporre la solita ricetta trita e ritrita, fatta di finanziamenti non strutturali, insufficienti, parziali, preferendo riproporre quanto è già stato fatto, e male, visti i costanti fallimenti dei provvedimenti emanati per il Mezzogiorno, e non abbia avuto - mi stupisce - il coraggio necessario per osare, ovvero

Signor Presidente, è all'esame dell'Assemblea la definizione dei criteri del costo *standard* per studente. Per restituire però la parola al Parlamento, c'è voluta la Corte costituzionale, che ha annullato i decreti con i quali i Governi passati si erano impossessati illegittimamente della competenza negli ultimi quattro anni. La ritrovata potestà legislativa ha consentito di emendare il testo per correggere almeno gli errori più gravi del metodo di calcolo. Il primo errore consiste nel calcolare il fabbisogno degli atenei escludendo il conteggio degli studenti fuori corso. Il criterio svantaggia gli atenei meridionali che ne hanno un numero maggiore. Con l'approvazione, però, dell'emendamento 12.25 si amplia il calcolo ai fuori corso di un anno, perché si tratta di solito di studenti che continuano a frequentare i corsi e spesso devono solo completare la laurea. Secondo punto: sommando i fabbisogni di tutti gli atenei si ottiene il fabbisogno totale del sistema universitario, che però non è mai stato utilizzato come parametro di riferimento negli anni passati. cioè, il Ministero ha applicato il costo *standard* agli atenei, ma non a se stesso. Non è casuale. Se si considerasse il fabbisogno totale, il finanziamento del sistema universitario dovrebbe aumentare del 20-30 Con l'emendamento 12.27 si obbliga il Governo a certificare il fabbisogno totale, che ogni anno sarà il punto di riferimento nella discussione sugli stanziamenti della legge di stabilità. Il terzo errore è il più grave. Il modello di calcolo vigente fa a cazzotti con la realtà. Consideriamo un semplice esempio tra due atenei che offrono due corsi: il primo con cento studenti e il secondo con cinquanta studenti. Il primo ateneo riceve un finanziamento doppio rispetto al secondo, pur affrontando entrambi gli stessi costi perché hanno gli stessi docenti. È evidente che il modello nasconde una grave distorsione dimensionale priva di qualsiasi giustificazione relativa ai costi reali. L'algoritmo determina, quindi, una forte penalizzazione degli atenei collocati in bacini poco attrattivi, meno accessibili o, comunque, a domanda più debole, soprattutto nelle università del Mezzogiorno, nelle aree interne del Centro e perfino in alcune Province del Nord, come in Liguria e in Friuli. Nei quattro anni passati molte risorse pubbliche sono state distribuite secondo criteri sbagliati e ingiusti, e viene da pensare che abbiano contribuito al calo delle immatricolazioni, che infatti è maggiore in quelle parti del Paese. Queste politiche sono inammissibili in un Paese come il nostro con una quota di laureati pari alla metà della media europea. Se si vuole davvero recuperare il ritardo occorre un balzo in avanti, una crescita dell'alta formazione per le nuove generazioni. non basta che l'università cresca nelle grandi città, ma si deve innalzare la qualità degli atenei nelle reti capillari del Paese, nella Provincia e tra gli strati sociali più svantaggiati. La correzione dell'algoritmo è ottenuta con l'emendamento 12.8 che determina la costanza l'emendamento 12.8 che determina la costanza del fabbisogno per numero di studenti, compreso tra valori minimi e massimi. In questo modo si rispecchia il funzionamento reale del sistema. Ovviamente, l'ateneo più grande sarà finanziato di più nella misura in cui offrirà un maggior numero di corsi, tenendo conto quindi dei suoi maggiori costi reali. Quarto errore: quando il numero degli studenti supera un numero massimo, il decreto sull'accreditamento dei corsi impone di aumentare quota parte del numero dei docenti, ma contemporaneamente un altro decreto, quello sul *turnover*, può impedire l'assunzione dei docenti previsti. nella situazione imbarazzante di non poter assumere il docente per il quale ha ricevuto un finanziamento aggiuntivo in base al costo *standard*. Siamo dentro un tipico comma in cui si affastellano regole che rispondono a logiche diverse. La coesistenza di algoritmi conflittuali determina contraddizioni e suscita comportamenti degli atenei non positivi per il sistema. L'effetto più negativo è la proliferazione del numero chiuso. Per evitare il doppio vincolo di dover aumentare docenti senza poterli assumere, l'ateneo fissa il numero chiuso al livello del numero massimo di studenti. Questa regolazione sarebbe inaccettabile nel sistema scolastico, che risponde, invece, alla crescita della popolazione studentesca con un corrispondente aumento del numero degli insegnanti. La stessa dinamica di sviluppo si dovrebbe verificare nell'università, se il Ministero applicasse coerentemente la logica del costo *standard*. Abbiamo cercato di liberare l'università da questo vincolo assurdo presentando l'emendamento 12.28, che elimina la norma Tremonti del massimale nazionale di *turnover*. *turnover*. Purtroppo, nonostante il testo fosse stato concordato con il MIUR, è stato bocciato dalla Commissione bilancio sulla base del parere negativo del MEF, privo a mio avviso di fondamento giuridico e contabile. Spero che in Assemblea si possa riesaminare l'emendamento. Con l'introduzione del costo *standard*, infatti, non ha più alcun senso il vincolo del *turnover*. Nel nuovo schema, infatti, la politica delle assunzioni degli atenei non può in nessun modo influire sulla crescita della spesa poiché è costretta a muoversi all'interno del *budget* assegnato con la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. il vincolo del *turnover* non serve a impedire la crescita del debito, vieta le assunzioni anche agli atenei che hanno risorse proprie, distorce la logica del costo *standard*. Eppure, questo vincolo ha danneggiato pesantemente l'università italiana, tenendo fuori dalla porta due generazioni di giovani studiosi, e causando un pernicioso invecchiamento della docenza. In conclusione, gli emendamenti del Gruppo PD, concordati con la ministra Fedeli, consentono di apportare importanti correttivi al modello applicato negli anni passati. Rimangono però altri problemi irrisolti: l'insufficiente finanziamento del fabbisogno totale, lo squilibrio a discapito dell'area umanistica - sociale, la mancata revisione generale delle regole di finanziamento dell'università. A tal fine, avevo proposto di limitare l'attuale decreto-legge all'inevitabile sanatoria dei quattro anni passati e di prevedere, invece, un altro disegno di legge per impostare su basi nuove un modello di finanziamento

del decreto-legge, senza una revisione generale della legge di finanziamento dell'università. Ormai tale esigenza è ineludibile. È necessaria una discussione pubblica e una riforma generale delle regole del sistema. Da dieci anni la politica universitaria è in balia di algoritmi apparentemente neutrali, inesorabili come le calamità naturali, incomprensibili ai non addetti ai lavori e inaccessibili al dibattito pubblico. Se ne sono serviti i Governi degli ultimi dieci anni per attuare la più pesante recessione nella storia del sistema universitario italiano, di triplice arretramento: circa il 20 per cento in meno di docenti, di fondi e di studenti. Nessun altro comparto della pubblica amministrazione ha subito un salasso di questa portata e nessun altro Paese europeo ha risposto alla crisi indebolendo così pesantemente le strutture dell'alta formazione e della ricerca. Esprimo in conclusione la soddisfazione per le utili correzioni introdotte nel decreto. Nei prossimi mesi, però, dovremo fare di più per apportare una correzione all'intera politica universitaria dell'ultimo decennio. Basta con il blocco delle assunzioni e con i numeri chiusi: bisogna aprire le porte dell'università ai giovani, ai ricercatori e agli studenti. È nel primario interesse del Paese.

su questo provvedimento ce la siamo posta. Ci siamo posti una domanda molto semplice, cioè se tutto va bene. La risposta è stata forse sì e forse no.

Credo, però, che sia stato un tentativo di rimettere in moto una parte di questo Paese che arranca faticosamente e che ha visto in questi ultimi anni di crisi il divario, non solamente con il Nord ma con la restante parte dell'Europa, aumentare

in legge del secondo decreto-legge che riguarda il Mezzogiorno emanato solamente quest'anno. Se poi dovessimo contare tutti i provvedimenti che, a vario titolo, si si sono susseguiti negli ultimi quaranta-cinquanta anni allora ci vorrebbe qualche giorno per metterli in fila. Se poi, signor Presidente, dovessimo relazionare sui risultati che tali provvedimenti hanno ottenuto, allora basterebbero probabilmente pochi minuti. al nostro esame si compone di 17 articoli che riguardano esclusivamente i territori del Sud, con diversi interventi in settori quali lo sviluppo imprenditoriale e industriale, l'agricoltura, l'agevolazione fiscale, l'occupazione, l'analfabetismo minorile e l'università, gli investimenti, l'ILVA e la marginalità sociale dovuta alla presenza degli immigrati.

Ho la sensazione che sia cominciata già da un po' di tempo la campagna elettorale e che si tenti di abbindolare il Meridione con qualche finanziamento, dato a pioggia, per garantirsi una certa visibilità. Sta di fatto che questo decreto-legge avrà lo stesso risultato di tanti altri provvedimenti, destinati a fallire per inconsistenza o per

Crisi e recessione hanno colpito l'intera economia mondiale in questi anni e hanno avuto un impatto pesante sul nostro sistema economico e ancor di più sulle Regioni meridionali, con effetto negativo su occupazione e redditi.

Forse è urgente che il Governo avvii un piano straordinario per il lavoro che viene invocato da tempo da più parti, indispensabile per far ripartire l'intero sistema economico in maniera strutturale e duratura.

un quadro in cui il Mezzogiorno è sempre più pericolosamente lontano dal resto del Paese e soprattutto dall'Europa. A tal proposito le politiche sino ad oggi adottate dal Governo non hanno certamente aiutato a migliorare la situazione del Sud,

Servono piani seri che possano riportare alla pari con altre aree europee un'area di questo Paese che ha sicuramente potenzialità enormi. Voi mi insegnate però che di potenzialità non si vive. Il rilancio per il Sud non può passare se non attraverso una riduzione delle tasse, ma questo deve valere per tutto il Paese e non può essere semplicemente

alcun piano industriale, ma l'ex presidente Renzi aveva presentato un *masterplan* per il Sud. Lo stesso *leader* dei giovani industriali chiedeva di coinvolgere nel

dell'articolo 11, recante «Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno»? È un bellissimo titolo. L'articolo è molto ben scritto, ma è poca cosa individuare aree di esclusione sociale per prevedere e promuovere progetti, altri tavoli e altre concertazioni che non servono a nulla e che probabilmente non porteranno da nessuna parte.

Calenda l'ha raccontata bene in Commissione e anche in tutte le riunioni che ha fatto con gli industriali: certo è che non abbiamo risolto grandi problemi. Signor Presidente, mai avrei avrei pensato che la crescita economica del Mezzogiorno potesse passare per l'azzeramento, attraverso un emendamento, dei rifiuti pericolosi. Tutto questo lo troviamo infilato nell'articolo 9 del provvedimento in esame, che magicamente fa uscire violette e margherite dai rifiuti, che solo poco prima erano considerati pericolosi.

Forse è il caso di ricordare il rapporto annuale sulle mafie e sui crimini ambientali. Forse lo sviluppo del Sud passa, invece, da una seria attenzione a queste enormi problematiche,

mi sono perso qualcosa per ciò che riguarda la questione industriale, ma forse il Sud dovrebbe concentrarsi su altre questioni, legate magari alla capacità di fare agricoltura e turismo. La proroga di un mese della misura agevolata, introdotta dalla legge di stabilità per il 2017, in materia di investimenti in beni materiali e strumentali ad alto contenuto tecnologico, potrebbe essere a tutti gli effetti una buona cosa, cosa, se non fosse che poi la gran parte di questi investimenti non viene fatta certamente al Sud. Non potevano certo mancare alcuni articoli sull'ILVA, eterno problema irrisolto, che ormai conta più commissari che operai. Speriamo che i soldi sequestrati alla famiglia Riva vengano effettivamente utilizzati per pagare i creditori e per la bonifica ambientale.

udite udite- sarà quello di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati. Potrei fare anche qualche nome della provincia di Bergamo, come la zona di Castione della Presolana

Presidente, mettiamoci anche la questione della valorizzazione dei terreni incolti e degli immobili inutilizzati e mettiamoci pure la creazione di Zone economiche speciali, per aumentare l'occupazione al Sud. però, in cuor mio, che l'idea del posto di lavoro pubblico debba essere un po' abbandonata e debba diventare meno attrattiva e che la società debba essere ben orientata a comprendere che il problema principale resta il lavoro, soprattutto quello femminile e giovanile. La soluzione è la compattezza e ci vuole serietà: non ci può essere responsabilità senza potere e non ci può essere potere senza responsabilità. Credo che di questo i nostri parlamentari del Sud dovranno sicuramente farne tesoro. L'approccio positivo verso la libera imprenditoria e verso la produzione deve essere estremamente serio.

mondo. La partenza o la ripartenza non possono non inglobare l'idea che bisogna passare dalle parole ai fatti,

non possa più funzionare come metafora: una locomotiva guida un treno in cui tutti i vagoni procedono alla stessa velocità. È vero, si fanno trainare, ma hanno la stessa velocità della locomotiva.

che aiuti loro a pensare che si può fare impresa nell'assoluta legalità, stando fuori da questioni legate a rapporti con mafia e via dicendo. Questo decreto-legge, probabilmente, scontenta un po' tutti: quelli del Nord si lamentano perché non hanno avuto qualche attenzione;

pensava di arrivare a un risultato del genere, credo che sia un pannicello caldo. Se l'idea è che possa innescare un meccanismo per cui

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 91 del 2017, recante disposizioni per la crescita economica nel Mezzogiorno, contiene talune misure sociali, ma è privo di una strategia progettuale sul Mezzogiorno. Innanzitutto c'è una prima grande perplessità che riguarda la necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla legge d'attuazione costituzionale n. 400 del 1988. Come è noto, questi principi sono stati ribaditi in diverse pronunce della Corte costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte ha osservato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto

Valutazione fatta sotto la propria responsabilità e sottoposta a giudizio del Capo dello Stato in sede di emanazione. La Corte conclude affermando che la necessaria omogeneità del decreto-legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione, riservandosi la facoltà di annullare le disposizioni introdotte dal Parlamento in violazione dei suindicati criteri. In alcuni casi nel testo in esame osserviamo un vero e proprio assalto alla diligenza, secondo una vecchia maniera. La proposta che prova a salvare la romanissima Accademia nazionale di Santa Cecilia, l'emendamento che tutela le condizioni di lavoro degli autisti dei camion, le deroghe per la formazione delle classi di alunni per le scuole danneggiate dal sisma nel Centro Italia, al di là del merito, che può essere perfino condivisibile, cosa c'entrano con lo sviluppo del Mezzogiorno? Vi sono poi tante stranezze: in tema di contrasto agli incendi boschivi, anziché introdurre una discutibile disposizione, che novella un articolo del codice penale dentro un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, perché non si è scelto di rendere operativa la legge n. 353 del 2000 che, per rafforzare la prevenzione, ha introdotto il catasto delle aree percorse dal fuoco, al fine di poter escludere queste aree da qualunque successivo progetto speculativo? Eppure oggi, a distanza di diciassette anni, i Comuni sono molto indietro, con la conseguenza che i vincoli del caso non possono essere applicati. se si può introdurre con assoluta leggerezza una norma che prolunga la permanenza in servizio dei magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 Per stare al merito del provvedimento, il testo che stiamo esaminando propone qualche pannicello caldo, ma nessun intervento strutturale e incisivo: in sintesi potremmo dire che non fa danni, ma è acqua fresca. Certo, possiamo sostenere che l'individuazione della misura a favore dei giovani nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» contiene propositi condivisibili, così come assume un valore senz'altro positivo l'approvazione in 5a Commissione di un emendamento del Gruppo Articolo 1-MDP che per questa specifica previsione innalza a 50.000 euro l'erogazione del finanziamento per ogni singolo richiedente che intende costituirsi in forma di impresa individuale o di società. Si continua però a percorrere una linea non risolutiva e cosi assistiamo perfino a vicende paradossali, come l'introduzione della norma che interviene sui consorzi agrari, con un'autentica forzatura che lede il principio di libera concorrenza, creando confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico, come sostenuto da diverse associazioni di settore. ora ad esporre sinteticamente alcuni indirizzi che si potrebbero adottare; sono solo esempi di un modo diverso di pensare al Mezzogiorno. Anzitutto occorre unire imprese e tecnologia sulla base di un disegno governato: solo con una regia istituzionale si possono far incontrare le piccole e medie imprese con la tecnologia. Si deve partire dalla consapevolezza che spesso le piccole imprese non sono in grado di esprimere e di formulare la domanda di innovazione a loro idonea (che rimane conseguentemente inespressa), pur sentendone genericamente l'esigenza. Più che di incentivi, l'ausilio alle piccole e medie imprese sul piano del progresso dei processi di lavoro necessita di una guida politico-istituzionale che si irradi in varie direzioni. Occorre creare un'interfaccia tra ricerca e impresa e puntare su figure intermedie di centri e professionisti che conoscano le problematiche della produzione e sappiano dialogare col mondo della ricerca applicata, per adattarla a ogni caso specifico, traducendola in progetti. Le imprese devono individuare facilmente il loro interlocutore dedicato o trovare sul mercato un'offerta privata di tali servizi ed essere incentivate a farlo. Le Regioni sono le prime indiziate per dedicare proprie istituzioni a questo compito. Buone iniziative in questo senso esistono già ma sono poche, concentrate prevalentemente al Nord e generalmente fanno capo alle camere di commercio. Il progetto allo studio del Governo di prevedere agevolazioni fiscali per l'impiego nelle piccole e medie imprese *digital angel* (esperti per l'abilitazione tecnologica) è meglio di niente, ma salta a piè pari la necessità di concepire una *governance* dei processi, che non si innescano da soli. Abbiamo bisogno nel Paese di almeno sei o sette centri di ricerca applicata a servizio delle imprese e come interfaccia delle lauree professionalizzanti. Si può cominciare dal Mezzogiorno per istituirli. Altro aspetto fondamentale è la logistica. Logistica e trasporti sono connessi anche con la questione meridionale. Dopo il raddoppio del Canale di Suez, il Meridione d'Italia dovrebbe proporsi come attrattore dei traffici mondiali che transitano nel Mediterraneo (20 per cento di tutti i traffici mondiali via nave) e connettersi al Nord con la Rete centrale nazionale (multimediale). Oggi il Sud risulta isolato dalle direttrici più importanti. L'alta velocità dovrebbe arrivare a Reggio Calabria e comprendere la Napoli-Bari-Taranto (che forse avrà un primo finanziamento nel 2017). Per ciò che riguarda il traffico crocieristico (per il quale siamo secondi in Europa, con 10 milioni di presenze), le Regioni andrebbero aiutate con cofinanziamenti a connettere il potenziamento del sistema portuale (e dei collegamenti con i porti) all'offerta sia turistica che produttiva del territorio retrostante, in un approccio integrato. Si dovrebbero stimolare le Regioni affinché i porti di approdo vengano trasformati in sé in punti di attrazione turistica e diventino parte integrante della vita sociale del tessuto urbano, con strutture ricreative, sportive e commerciali e con rigenerazione paesaggistica. La rete ferroviaria nazionale e regionale dovrebbe essere unica e integrata, capace di soddisfare le interconnessioni rilevanti. Poi c'è la questione delle reti d'impresa. Possono andare dall'aggregazione per lo sviluppo del territorio alla messa in comune di servizi *post*-vendita in qualche parte del mondo o di un *export manager*, allo sviluppo comune di progetti di ingegneria. Occorre puntare con più determinazione su queste aggregazioni: non sono sufficienti i 122 milioni spesi negli ultimi cinque anni in questo tipo di progetti. Occorre riprendere l'impegno nazionale di detassazione di quanto le imprese destinano al patrimonio delle reti per iniziative comuni (solo 9 milioni per le reti di impresa per l'artigianato digitale e 8 milioni per le reti di impresa operanti nel turismo, con clausole restrittive). Quanto all'università, si è puntato su sporadiche eccellenze, in un quadro medio non eccelso, piuttosto che a elevare la qualità media generale, con la conseguenza di produrre una differenziazione fortissima tra sedi, che è anche territoriale. Questo ha penalizzato le università del Sud. È mancato un impegno sulle università, i cui docenti sono passati da 62.000 nel 2008 a 50.000 nel 2016, da oltre 320.000 a meno di 260.000, con un taglio di fondi del 20 per cento. Si registra anche una migrazione di studenti dal Sud al Nord, non sempre giustificata dalla qualità dell'offerta formativa, ma solo dall'aspettativa di migliori opportunità occupazionali. Assegnare i fondi solo per il 28 per cento su base delle iscrizioni e il resto su base premiale vuol dire penalizzare le università del Sud. L'università è stata lasciata a sé stessa e senza scenari di domanda formativa piuttosto che farne elemento della crescita del Paese. Molti meccanismi sono perversi: allocazione dei fondi, selezione e sostituzione dei docenti, processi di valutazione, assenza di piani di riequilibrio basati su patti e verifiche (indispensabili per il Sud), tipologie delle offerte formative, organizzazione della ricerca, concorrenza invece che collaborazione. Occorre una revisione. Le lauree di primo livello non hanno raggiunto lo scopo, se il 55 per cento dei laureati prosegue per le lauree magistrali (cinque anni di media per le lauree triennali, con 1/3 con voti bassi, inferiori a 90). A cinque anni dalla laurea, solo il 50 per cento utilizza pienamente le competenze acquisite. Il «tre più

i percorsi di studio brevi più direttamente legati alle professioni tecniche di livello alto. Sono necessarie lauree professionalizzanti con un anno di teoria, uno di laboratorio e uno di formazione sul lavoro; vanno istituite e incardinate nelle università. In Germania producono tra il 30 e il 40 per cento dei laureati. La conferenza dei rettori si sta ponendo il problema, la nostra classe politica no. Senza un'istruzione tecnica applicata sarà difficile per la nostra industria prosperare. L'apprendistato di alta formazione non decolla. Non possiamo lasciare il problema agli istituti tecnici superiori, che sono solo 74. Ci vuole una *governance* di questi processi, soprattutto nel Sud. Per il diritto allo studio occorre una regia unitaria che coordini l'impegno regionale e nazionale (il fondo integrativo è stato decurtato dopo il 2008 e solo ora è in risalita), evitando sperequazioni che fanno sì che al Nord ricevano la borsa il 90 per cento degli idonei e al Sud il 50 per cento. Sarebbe necessario assorbire nella responsabilità pubblica quanto cade sugli atenei in termini di minori introiti per gli sgravi alle tasse universitarie. Occorre incrementare gli investimenti per residenze universitarie. Signor Presidente, colleghi, anche se l'ultimissimo dato rileva nel Sud una ripresa al pari di quella dell'Italia intera, devono essere tenuti presenti gli effetti dell'austerità dal 2008, che sono stati più profondi nel Sud per diminuzione del reddito, per occupati, per calo degli investimenti pubblici, per disinvestimento nelle università,

Il *masterplan* per il Sud, nell'ambito del quale vengono siglati patti con le Regioni e con alcune città del Sud, porta alla frammentazione dei progetti. Si tratta di una ricognizione delle risorse esistenti, dell'elenco degli interventi da attuare, con data e spesa. Va apprezzato che questi patti ci siano ed è un passo avanti, ma nella sostanza siamo di fronte solo a un tentativo di accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali e a una sostanziale riproposizione di progetti dormienti, su cui confluiscono in modo tardivo e parziale risorse già destinate al Sud. Non vi sono impegni aggiuntivi rispetto all'ordinaria spesa pubblica (assegnazione di 13,3 miliardi deliberati dal CIPE sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, che stanziava per il Sud 44 miliardi per il periodo 2014-20; gli altri saranno sbloccati con decisioni del CIPE solo dal 2018). La progettazione dei fondi rimane piena di duplicazioni. In conclusione, è un'illusione continuare a pensare che lo sviluppo possa salire dal basso verso l'alto. Occorre un soggetto che produca un coordinamento di sistema, che organizzi capitali e soggetti privati e pubblici, interagisca con i territori, svolga politiche di attrazione degli investimenti legate all'unicità degli stessi, interagisca con i distretti tecnologici e industriali e con le città; soprattutto, che stabilisca le priorità. Non un soggetto che gestisca denaro, ma che coordini e indirizzi, cercando di accompagnare il cambiamento. Inoltre, in assenza di investimenti pubblici che aggrediscano le condizioni di sottosviluppo di intere aree del Sud, creando occupazione stabile e qualificata, il rischio serio è che, dopo alcuni *slogan* evocativi, i risultati continueranno ad essere insufficienti. *(Applausi

l'intero territorio del basso Molise è stato messo in ginocchio da un devastante incendio che ha determinato la chiusura dell'autostrada A1 nei due sensi di marcia, della linea ferroviaria adriatica e della strada statale 87, spaccando il Paese in due per tutto il pomeriggio della giornata di ieri. Tutto il pomeriggio le istituzioni sono state assenti. Il sito della Regione non ha dato alcun comunicato sui fatti. Il sito della Protezione civile, che era fermo al 7 luglio di quest'anno, è stato aggiornato soltanto nella tarda serata di ieri. Praticamente, un intero territorio della Regione Molise è stato lasciato solo, senza che le istituzioni intervenissero. È venuto meno, in questo modo, il coordinamento delle operazioni, con gravi ritardi nello spegnimento dell'incendio e con gravissimi rischi a carico della popolazione. Sono state lambite dalle fiamme le case sia nel Comune di Termoli, sia nel Comune di Guglionesi ed è stata persino evacuata la fabbrica della FIAT, dove lavorano 4.500 persone.

finestra"), alla quale non ho avuto ancora risposta. Prego questa Presidenza di attivarsi perché il Governo risponda alla mia interrogazione. Signor Presidente, approfitto della presenza di un Ministro e di un Sottosegretario per far presente una questione che preoccupa letteralmente tutta la popolazione trentina. Circa una ventina d'anni fa, l'Unione europea aveva proposto al Ministero dell'ambiente l'introduzione dell'orso in alcuni territori, il famoso progetto Life Ursus sono state introdotte, in più sequenze, coppie di orsi provenienti dalla Slovenia. Adesso il problema diventa grave: oggi stesso ci sono persone in ospedale in condizioni abbastanza gravi. Negli ultimi tre anni si sono verificati quattro episodi che hanno comportato lesioni importanti e ricoveri ospedalieri: a Pinzolo, in prossimità delle funivie di risalita;

con il proprio cane; tre giorni fa è successo più o meno nelle stesse zone, a Terlago, dove una persona è viva per miracolo, con lesioni alle gambe e alle braccia, ma se l'è cavata perché aveva un cane, che ha disturbato l'orso e pertanto la persona è riuscita a svincolarsi. Chi sono e dove sono? Non tutti gli orsi hanno un radiocollare, per cui non si riesce nemmeno a localizzarli. Diciamo che questo progetto non è stato ben gestito.

Di trovare una soluzione, in sintonia con la Provincia autonoma di Trento, che ha in parte le mani legate. Bisogna stabilire che adesso gli orsi - che sono indubbiamente in sovrannumero - rappresentano un problema di incolumità pubblica.

possibilità e la capacità di gestirli si prospetta un problema di incolumità pubblica. Signor Presidente, dieci anni fa un vasto incendio deturpò Peschici, distruggendo centinaia di ettari di bosco, con un drammatico bilancio di tre morti e decine di feriti. Ieri, sempre a Peschici, nel Parco nazionale del Gargano, nella baia di Manaccora, il fuoco è tornato a seminare distruzione. Tantissime sono le case interessate dall'incendio. A causa delle fiamme è stato bloccato anche il tratto della strada statale 89, in località Mandrione, per evitare ulteriori disagi per gli automobilisti in transito. Come se non bastasse, l'incendio ha continuato la sua opera di devastazione per tutta la notte, proprio tra Peschici e Vieste, polverizzando la macchia mediterranea circostante, con danni incalcolabili per l'ecosistema e l'ambiente. Il Gargano, dunque, torna a essere lo scenario di eventi causati da piromani e gente senza scrupoli, dopo essere già stato vittima, in passato, di altri incendi. altresì la ferita, ancora aperta, relativa al settembre 2014, quando fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità hanno causato gravissimi danni: è vergognoso che per un evento risalente a tre anni fa siamo ancora a chiedere quale sia lo stato di ottemperamento degli interventi previsti e di avanzamento e cantierizzazione dei lavori.

Approfitto per dire che il Gargano non deve essere lasciato solo, ma deve essere tutelato e sorretto dallo Stato. Soprattutto, bisogna evitare che si verifichino ancora questi episodi

Signor Presidente, colleghi senatori, il mio intervento oggi, a fine seduta, prosegue la staffetta attraverso cui, insieme a tante senatrici e senatori, ormai da più di un anno, abbiamo deciso di ricordare ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da una relazione sentimentale. Continueremo con questa staffetta fino a quando sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. In poco più di un mese, altri due delitti si sono aggiunti alla lunghissima catena. Mi riferisco a Erika Preti, una ragazza di ventotto anni, di Pralungo, in provincia di Biella, è stata uccisa l'11 giugno scorso mentre si trovava in vacanza in Sardegna con il fidanzato, il quale, dopo aver addebitato per settimane la responsabilità a un fantomatico rapinatore, solo due giorni fa ha confessato di essere il vero autore del delitto. Ciò che rende ancora più drammatica, se possibile, la scomparsa di Erika è la motivazione che avrebbe scatenato l'intenzione omicida del fidanzato, cioè l'essere stato rimproverato da lei per delle briciole di pane sul tavolo. E ancora, il 24 luglio, a Musile di Piave, in provincia di Venezia, Maria Archetta Mennella, di 38 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex marito,

Da ultimo, appena ieri, a Castellammare c'è stato un femminicidio per fortuna solo tentato: un incontro tra due ex fidanzati, che doveva essere rappacificatore e che si è concluso con l'uomo che ha brutalmente investito con la sua auto la donna condizioni, è riuscita a chiamare direttamente i soccorsi. Con questi episodi, salgono a 71 le donne che abbiamo ricordato in questa staffetta, iniziata nel 2016. I dati presentati dall'ISTAT a fine marzo scorso sulla violenza di genere ci confermano che il femminicidio è solo la conclusione più estrema di un diffuso problema di violenza maschile sulle donne quei dati sono impressionanti: 8 milioni sarebbero le donne vittime di violenza psicologica, 4,5 milioni le donne che hanno subito nell'arco della propria vita atti sessuali degradanti ed umilianti, rapporti subiti con violenza, abusi, tentativi di stupro e stupri. Signor Presidente, con queste testimonianze riproponiamo con convinzione il nostro appello, un appello innanzitutto al Governo ed in particolare alla Sottosegretaria con delega alle pari opportunità: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi ed i limiti della legge n. 119 del 2013

perché si rischia di colpevolizzare le donne che invece della violenza sono vittime ed al Paese intero diciamo che non si può accettare da nessun punto di vista che nel solo ultimo anno siano un centinaio le donne uccise nel nostro Paese con modalità e motivazioni simili In conclusione, mi sembra appropriato citare una frase che Maria Archetta Mennella ha scritto in un *social* qualche giorno prima di essere uccisa, una frase che mi sembra un monito rivolto alla qualità dei rapporti di genere: «Mi fanno paura» -scriveva la donna - «gli uomini che non capiscono che amare qualcuno vuol dire amare la sua libertà».